La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità di inserire quale unico punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani la discussione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo collegato alla Convenzione quadro ONU

dai provvedimenti non conclusi (collegato lavoro autonomo, mozioni sull'adeguamento delle infrastrutture idriche e disegno di legge su parchi e aree protette). Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 novembre si svolgerà il *question time* con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Infine, su richiesta del Gruppo Lega Nord, la seduta pomeridiana di oggi terminerà alle ore 18,30.

Prendiamo atto della disponibilità, assunta dalla maggioranza già in Commissione, a recepire i suggerimenti ed i consigli pervenuti da larga parte dell'Assemblea; prendiamo atto della volontà del relatore Martini e del

prendiamo atto che il Governo si impegna anche a rivedere la procedura e la normativa in tema di dichiarazioni

dichiarazione della condizione di monumento nazionale. Effettivamente, si riscontra che per questo tipo di provvedimenti estremamente semplici l'Assemblea e le Commissioni vengono impegnate in maniera troppo dispersiva.

la figura di Gramsci, intellettuale eclettico e dinamico, politico lungimirante, ma soprattutto scrittore di straordinaria intelligenza, ha contribuito a sviluppare la coscienza critica del Novecento. Antonio Gramsci è stato senza dubbio un uomo di spicco della cultura sarda e italiana. Persona seria, profondamente onesta che, come Emilio Lussu, anch'egli grande combattente politico, ha saputo esprimere al meglio nell'arco della sua breve vita l'attaccamento orgoglioso alla Sardegna e alle sue origini. Tuttavia, nonostante il grande rispetto che è naturalmente e necessariamente dovuto a un pensatore di questo calibro, riteniamo che il disegno di legge che oggi ci vede impegnati in quest'Aula abbia diverse opacità, che non possiamo ignorare nonostante tutto. Il nostro ordinamento non prevede una definizione di monumento nazionale né, pertanto, alcuna disciplina applicabile. La conseguenza è che, con l'approvazione di questo provvedimento, non si avrebbe la produzione di alcun effetto giuridico, salvo l'attribuzione di una mera onorificenza. La mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo non può sconfinare nella violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Ne deriva che, quando eccezionalmente l'attività legislativa è volta alla realizzazione di attività di carattere non generale ed astratto, bensì particolare e concreto, devono sussistere validi motivi e si devono conoscere i criteri in relazione ai quali sono effettuate effettuate le scelte e le relative modalità di attuazione. Nel ribadire il grande rispetto e, nel mio caso, in quanto sarda, il particolare attaccamento a questa figura, simbolo della Sardegna e del mondo, vogliamo scongiurare che questa occasione crei privilegi che comportino erogazioni di fondi pubblici a favore di un sito culturale e a discapito di altri. Si tratta solo di una questione di metodo e di sostanza. Siamo certi Siamo certi che la Casa Museo di Antonio Gramsci non possa essere tutelata, valorizzata e protetta con gli strumenti legislativi già esistenti? Sarebbe più ragionevole operare una scelta basata sull'individuazione di una definizione aggiornata di monumento nazionale nell'alveo di un quadro normativo coerente. Sarebbe importante novellare il codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di statuire nuovi e adeguati parametri. Ci sembra corretto non adottare leggi provvedimento fin quando non si arrivi alla definizione di un quadro normativo in cui il significato di monumento nazionale sia chiaro e preciso. Per questi motivi, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario, proprio perché non siamo indifferenti alla cultura e vorremmo soprattutto che la Casa Museo, che è luogo di conoscenza, non versasse nella situazione di abbandono nella quale si trova ora.

la mia dichiarazione sarà un po' più lunga rispetto a quelle che mi hanno preceduto, perché il mio Gruppo non è intervenuto in discussione generale. Oggi il Senato è chiamato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di legge avente ad oggetto la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci di Ghilarza. È il luogo dove, tra il 1898 ed il 1914, visse Antonio Gramsci, sardo nativo di Ales, uno dei maggiori intellettuali del nostro Novecento. Di Antonio Gramsci è molto conosciuta la storia politica: è stato tra l'altro, nel 1921, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. Ma lo stesso si occupò a tutto campo anche filosofia, di storia, di letteratura, di glottologia, di teatro e di tradizioni popolari, esplorando con passione e competenza diversi ambiti della conoscenza. Gramsci è l'autore italiano del Novecento tradotto in più lingue: non dispongo di elementi statistici per verificare l'affermazione, ma è certo che i suoi scritti sono studiati più all'estero che in Italia, dove forse è prevalsa sinora una lettura quasi esclusivamente politica e di parte del grande pensatore. Intendiamoci, Gramsci era un uomo di parte, ma al tempo stesso esprimeva una personalità complessa, che richiede ancora oggi adeguati studi e approfondimenti:

e sulla sua vicenda carceraria (penso in particolare agli scritti di Luciano Canfora e Franco Lo Piparo) ha posto in luce nuovi elementi di riflessione e interrogativi cruciali, che riaprono i termini di una discussione sempre attuale. Gramsci è dunque un personaggio studiato, molto studiato, ma ancora da scoprire. La Casa Museo che per legge dello Stato deve diventare monumento nazionale è la casa sita a Ghilarza, centro dell'Alto Oristanese che insiste su un pianoro vulcanico, dove Gramsci, a partire dal 1898, visse con la sua famiglia d'origine gli anni della seconda infanzia e dell'adolescenza. È sicuramente un luogo della memoria di interesse nazionale (e non solo) perché rappresenta lo spazio fisico nel quale le vicende personali di Gramsci si sono intrecciate, negli anni della sua formazione, con quelle della storia d'Italia. Ed è questa la ragione principale per la quale la Casa Museo Gramsci verrà dichiarata monumento nazionale. Sono pertanto ravvisabili una molteplicità di ragioni storiche, culturali e politiche che giustificano la dichiarazione di monumento nazionale da parte del Parlamento. È stato obiettato - e mi riferisco al voto contrario annunciato dal Movimento 5 Stelle - che nel nostro ordinamento non esiste alcuna definizione di monumento nazionale, per cui staremmo approvando un qualcosa che non esiste. Ora, a prescindere dalla considerazione che, nella formazione degli ordinamenti giuridici democratici il diritto è sempre preceduto dal fatto, essendo il legislatore chiamato a dare una disciplina a ciò che esiste, è semplice osservare che, in politica, il valore simbolico è sempre molto forte e denso di significati. La dichiarazione di monumento nazionale, che il Parlamento si accinge ad approvare, tra l'altro, fa seguito al decreto decreto del 26 gennaio 2016, n. 16, adottato dalla competente Soprintendenza alle belle arti e del paesaggio, che ha dichiarato la Casa Museo Gramsci bene d'interesse storico, culturale ed artistico ai sensi del codice dei beni culturali. Ma si tratta di due cose diverse, ancorché in parte convergenti, posto che la Soprintendenza impone un vincolo storico-artistico basato su un giudizio di natura tecnica e non politica. Qui il valore simbolico - come è stato osservato anche da altre parti - risiede nel riconoscimento della grande valenza storica del pensiero e dell'azione di una delle più importanti figure del Novecento. Tale passaggio non significa che l'opera dell'intellettuale sardo debba essere necessariamente condivisa da ciascuno di noi e in tutti aspetti. Ciò che non può essere disconosciuto è la grandezza dell'uomo e il suo contributo alla formazione della cultura nazionale, così come i socialisti o i liberali, tanto per fare un esempio, riconoscono la grandezza di don Sturzo o di De Gasperi o, ancora, ciascuno di noi riconosce l'importanza di Benedetto Croce ancorché, in ipotesi, non condivida l'idealismo crociano. Affermare che «Gramsci è di tutti» significa riconoscere il valore di una persona che ha dato un contributo originale alla costruzione di una cultura nazionale, quella italiana,

non può essere circoscritta al patrimonio di un singolo partito politico (e, con tutta onestà, oggi non saprei dire quale) ma deve entrare a far parte, a pieno titolo, della storia civile del nostro Paese e della cultura internazionale, fatto che, come ho detto, documentato dalle numerose traduzioni delle sue opere nelle principali lingue del mondo. Di fronte a personalità di tale spessore, costituisce un giusto riconoscimento attribuire un rango specifico e simbolico al luogo fisico nel quale le stesse mossero mossero i primi passi e lasciarono durevoli tracce di affetti. In questa prospettiva, la modesta casa dei Gramsci, costruita in pietra lavica nel centro storico di Ghilarza, rappresenta il punto d'inizio di una vicenda esistenziale che ha lasciato il segno, ben oltre ed al di là della sua durata effettiva. Voglio anche evidenziare il forte legame di Gramsci con la Sardegna e con Ghilarza in particolare: un legame denso di significati che attraversa in profondità tutta la sua vita e la sua opera e che troviamo fortemente presente sopratutto nelle «Lettere dal carcere» che, segnando gli affetti più intimi, racchiudono forse l'espressione più nitida della sua complessa personalità. Penso che dobbiamo essere grati a quanti, nel corso degli anni, hanno consentito che questo importante patrimonio non venisse disperso e cancellato dalla memoria collettiva:

Auspico infine che, superato ogni conflitto (proprio nei giorni scorsi il principale quotidiano della Sardegna, «L'Unione Sarda» ha dato notizia dello sfratto intimato alla Casa Museo), la proprietà Museo), la proprietà e la gestione del bene, per il rilievo che sempre più vengono ad assumere, siano affidati ad una gestione plurale, espressione delle istituzioni, delle associazioni e degli studiosi che maggiormente hanno dedicato il loro tempo e le loro energie all'analisi del pensiero di Gramsci senza spirito di parte.

con la pietra lavica, che è la pietra tipica di quel territorio. In quel territorio e in quella casa Antonio inizia la sua formazione scolastica e culturale. Dopo pochi anni, la sua famiglia, ridotta in condizioni di povertà, in particolare per l'assenza del padre, deve provvedere alle proprie necessità arrangiandosi come può e anche Antonio, che è il quarto di sette figli, pur avendo una grande passione per gli studi, non può iscriversi al ginnasio ed è costretto ad andare a lavorare, come lui stesso ricorderà, all'ufficio del catasto di Ghilarza, dieci ore al giorno per nove lire, che era il prezzo di un chilo di pane. Negli anni seguenti, egli riuscirà a riprendere gli studi e a concludere il liceo nel 1911. In quello stesso anno, grazie a una borsa di studio, riesce a iscriversi all'università di Torino. Nel 1911 Gramsci lascia per la prima volta la Sardegna e si trasferisce in una Torino industrializzata e in pieno fermento sociale e politico,

e la Sardegna, Ghilarza e la casa di famiglia faranno parte dei suoi ricordi di adulto, rappresenteranno le sue radici più profonde e saranno poi la lente con la quale penserà al mondo nei lunghi e duri anni di prigionia. Certo, quella casa non rappresenta l'unico luogo della formazione di Gramsci; molto hanno rappresentato per la sua formazione Torino, Roma, Mosca purtroppo, le diverse tappe che i carceri gli hanno imposto di fare, tuttavia la casa di Ghilarza, per certi versi, è stata per la sua intera esistenza l'unico luogo che Gramsci ha identificato veramente come la sua casa familiare. E, allora, perché fare della casa dei Gramsci un monumento nazionale? Non credo sia solo per rendere omaggio ad un uomo che ha pagato con il carcere e poi con la vita le sue convinzioni filosofiche e politiche. Credo, invece, sia corretto, a maggior ragione oggi, mantenere un giudizio il più possibile storico e completo della figura di Gramsci. Alla sua vicenda umana di uomo privato della propria libertà va sempre associata la sua natura principale di pensatore e di politico. È vero, da alcuni scritti giovanili e, ancora più, in quelli raccolti nei quaderni dal carcere, emerge un Gramsci appassionato di storia, curioso e appassionato della filosofia e della letteratura (come

a sua moglie Julca Schucht o ai suoi figli Delio e Giuliano; quando pensa alla sua famiglia e al suo paese.

scriverà più tardi: «Quante volte avrò detto "a mare i continentali"», che è a un'espressione che noi sardi conosciamo ancora molto bene per arrivare a guardare la Sardegna, seppure con le sue peculiarità, come ad un pezzo d'Italia. Tatiana: «Io stesso non ho alcuna razza. Mio padre è di origine albanese, tuttavia, la mia cultura è italiana, fondamentalmente questo è il mio mondo». mondo». Da una cella in cui è recluso dalla dittatura fascista, Gramsci riesce a pensare prepotentemente alla vita, alle persone e alle loro vicende. Forse si sofferma su quegli aspetti anche in maniera più attenta di come avrebbe fatto nella sua condizione di uomo libero. Certo, Gramsci era tutto questo e anche questo, oggi quelle «Lettere dal carcere» rappresentano un patrimonio per l'intera letteratura dell'umanità. Sicuramente già questo sarebbe sufficiente per rendere la sua casa dell'infanzia e dell'adolescenza monumento nazionale. Gramsci era, però, innanzi tutto, un ideologo, un politico, ed era soprattutto uno dei fondatori, nel 1921, del Partito Comunista Italiano. Né il carcere né la malattia hanno mai scalfito il suo convincimento della necessità di costruire una società nuova, un destino diverso per l'umanità, la liberazione di tutti gli oppressi e delle classi sociali subalterne dal giogo dello sfruttamento. Gramsci scriveva: «La Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio». È questo il pensiero di uno che era uomo di parte, un comunista. Centrale, poi, com'è noto, è la sua elaborazione sul concetto di egemonia, uno degli aspetti più studiati del pensiero gramsciano: le classi dominanti impongono i propri valori politici, culturali, la propria morale al resto della società; chi può imporre questi valori gestisce il potere e mantiene insieme classi dominanti e classi subalterne. In Gramsci il sogno di una nuova società di uguali si concilia sempre con l'idea di una società di liberi,

si interrogano sulla conciliabilità delle sue posizioni con quelle espresse da altri pensatori comunisti come lui, suoi contemporanei, ortodossi, quelli dopo la rivoluzione del 1917, alla linea marxista-leninista. A mio parere, non è solo l'articolazione di pensiero politico e filosofico, ma è, in particolare, la conciliazione del sogno di una nuova società, della partecipazione di intere masse al proprio destino e di libertà, che ha reso Gramsci il pensatore italiano del Novecento più studiato e letto nei cinque Continenti; anzi, ad oggi, uno degli italiani più conosciuti di tutti i tempi. La casa di Gramsci, che è divenuta negli anni Sessanta sede della omonima associazione, è stata un centro di rapporti tra ex partigiani, intellettuali, sindacalisti e studiosi, che furono i promotori, negli anni Ottanta, della sua restaurazione. Oggi è un museo e un centro di documentazione, di ricerca e di attività culturali. Se essa è meta di visitatori provenienti da tutto il mondo, e in particolare di giovani studenti, il merito è di tutti coloro che hanno cercato ostinatamente di mantenere quella casa come il luogo della memoria gramsciana, prima tra tutti la sorella Teresa, l'amatissima Teresina per Gramsci, e le sue due figlie Diddi e Mimma Paulesu. Che cosa resta oggi di Antonio Gramsci? Dopo la caduta dei muri e l'esperienza, inizialmente esaltante e poi drammatica, dei Paesi che aspiravano a fondarsi sui principi marxisti, resta un Gramsci vitale e centrale nel pensiero democratico moderno di diverse generazioni non solo italiane e in una dimensione planetaria. Dice giustamente l'economista premio Nobel, Amartya Sen, che l'influenza di Antonio Gramsci sulla storia della filosofia va molto al di là del marxismo. Con la casa di Gramsci monumento nazionale vogliamo ricordare a noi tutti e alle future generazioni un uomo, un pensatore, un politico e un pezzo di storia del nostro Paese che è giusto preservare qualunque sia il giudizio storico e politico che si voglia dare al suo pensiero. Vorrei ringraziare per l'iniziativa assunta dalla nostra collega, onorevole Pes,

Grazie Presidente, dal voto per ragioni di metodo e merito. La ragione di metodo riguarda l'uso o - meglio dire - l'abuso dello strumento legislativo, che non ritengo necessario per tutelare i molti simboli della nostra memoria. Dal punto di vista del merito, porto rispetto per la vita e il pensiero di Antonio Gramsci, che ritengo sia stato spesso originale e profondo, ma credo che non abbiamo una memoria condivisa dalla Nazione, come taluni hanno invece affermato oggi. Anzi, non abbiamo nemmeno una memoria condivisa dalla sinistra italiana.

Signora Presidente, giunge finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento atteso, collegato al disegno di legge di stabilità riferita all'anno in corso

a leggere alcune considerazioni di carattere generale, consegnando alla Presidenza la puntuale descrizione del provvedimento,

Il cambiamento del lavoro inizia ad essere finalmente compreso nella sua profondità. Le nuove tecnologie digitali hanno effetti pervasivi per cui ogni programma orientato a diffonderle, come il recente Industria 4.0 del Governo, non può prescindere dalla relazione biunivoca tra esse e il mercato del lavoro. Recentemente il World Economic Forum ha sottolineato come i principali cambiamenti sottesi alla grande trasformazione del lavoro si produrranno nei prossimi cinque anni e perciò richiedono una immediata strategia al fine di evitare polarizzazione dei benefici professionali e reddituali su un'esigua minoranza di lavoratori, disoccupazione di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale. Fattori demografici, inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università con particolare riguardo alla ricerca, nei servizi creditizi e finanziari, collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e agilità che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, cambiano il lavoro con caratteristiche di velocità e di imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e di servizi, di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization*, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride,

generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o nei modi di erogare servizi. Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su impresa e lavoro, non sono solo di tipo economico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, come diciamo da tempo, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono esse stesse, oggi, lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutate sulla base della produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'orario di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento del lavoro non sono più considerati in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità, insomma, diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative. Essa non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo, così come la migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia non è l'unico potenziale beneficio per il lavoratore. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti, immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Per questo le norme devono essere semplici e certe. Una *soft regulation*, come diceva Biagi, di tipo promozionale, con rinvio all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore delle modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. La libera contrattazione collettiva, soprattutto di prossimità, potrà sempre offrire una utile cornice. Necessario sarà però anche un piano straordinario di alfabetizzazione digitale, utilizzando i fondi interprofessionali, con lo scopo di riqualificare i molti lavoratori che in Italia sono stati a lungo occupati nelle attività ripetitive della tradizionale produzione manifatturiera e che devono ora transitare verso nuove professioni. In questo contesto, le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più ha vissuto processi di impoverimento relativo, e nel presente vivono una condizione di fragilità, accentuata dalla elevata pressione fiscale e regolatoria, nonché dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Non si tratta di partire dal presupposto che i titolari di partita IVA siano involontariamente tali e perciò aspiranti alla subordinazione, definendo in conseguenza le tutele, ma di individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli effetti negativi, attraverso forme di protezione compatibili con la natura autonoma, di essere soggetti ad una tassazione più equa e ad una regolazione semplice, di essere maggiormente protetti dalla legge nei rapporti contrattuali, di poter valorizzare le capacità professionali attraverso investimenti detassati nella continua riqualificazione delle proprie competenze, la possibilità di partecipare, anche in forma associata, ai bandi di gara e la stessa capacità, quando organizzate in ordini, di svolgere funzioni di pubblico interesse in una logica sussidiaria. Dobbiamo comunque considerare le possibilità di consolidamento e sviluppo tanto delle professioni ordinistiche, quanto di quelle non ordinistiche. Alcuni rilevanti profili, pure oggetto di esame in Commissione, sono stati poi rinviati alla legge di stabilità in ragione degli oneri che comportano. Ci si riferisce ad alcune misure in materia tributaria, come una definizione più certa della "autonoma organizzazione" ai fini del pagamento dell'IRAP o il definitivo superamento degli studi di settore, con modalità premiali dell'affidabilità fiscale, alla riduzione dell'aliquota previdenziale, al superamento o alla riorganizzazione in termini trasparenti della stessa gestione separata presso l'INPS, alla definizione certa della possibilità di partecipare dei Confidi e di avere le relative garanzie. modo si dovranno individuare modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali, per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa la equità della remunerazione. Mi avvio a concludere, citando Marco Biagi, il quale ci diceva, con preveggenza, che «la stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (...) appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani» così diceva allora «diventa un collaboratore che opera all'interno di un "ciclo". Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale». Pensate alle conseguenze sul piano dei versamenti contributivi, per cui non un euro di versamento contributivo può essere perduto in questa vita lavorativa così diversa da quella che abbiamo Ne deriverebbe quindi l'esigenza di uscire dal vecchio e pesante impianto regolatore del lavoro, figlio del vecchio mondo, attraverso un testo unico disegnato sul "suo" Statuto dei lavori, rivolto cioè a regolare in modo essenziale tutti i lavori con poche norme inderogabili fondate sui principi costituzionali e comunitari, tutele proporzionate alla effettiva fragilità socioeconomica in ogni tipo di prestazione e principalmente rivolte alla occupabilità, molto rinvio molto rinvio alla contrattazione di prossimità, anche individuale, o al rapporto specifico tra committente e prestatore per la reciproca adattabilità tra le parti. In attesa In attesa di una ambiziosa e duratura sintesi, quale appunto ho qui auspicato, quella di un testo unico denominato «Statuto dei lavori», la disciplina la disciplina del lavoro ha tuttavia bisogno di ulteriori misure urgenti per il sostegno alle libere professioni e lo sviluppo del lavoro "agile". che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è la sintesi del disegno di legge del Governo n. 2233, collegato alla legge di stabilità 2016, e del disegno di legge a mia prima firma n. 2229. 2229. La Commissione ha svolto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un buon lavoro di sintesi, in un clima che credo di poter definire cooperativo.

ad altri strumenti normativi gli ulteriori interventi che gli ordini del giorno potrebbero indicare. Ordini del giorno che potrebbero sostituire anche molti degli emendamenti proposti, per cui potrà valere la pena esaminarli al punto in cui li troveremo, per individuare, se condivisi (e molti di essi lo sono), luoghi nei quali trovare per essi una soluzione legislativa. annunciato, per il resto consegno una descrizione puntuale delle modifiche e delle integrazioni introdotte dalla Commissione e, più in generale, del testo che è all'esame dell'Aula e che, mi auguro, presto giungerà

Signora Presidente, negli ultimi decenni di fatto la richiesta di nuove figure professionali da parte del mercato, accompagnato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, di norme che hanno fatto nascere nuovi contratti di collaborazione, ha reso la categoria del lavoro autonomo molto diversa dal passato, e certamente non meno degna di protezione di quella del lavoro dipendente. Anzi, gli effetti della crisi economica degli ultimi anni si sono abbattuti su di essi e solo ultimamente si è accelerato il loro riconoscimento come categoria di lavoratori bisognosi di attenzioni e di tutele, anche per la debolezza, se non l'assenza, per molto tempo, di strumenti associativi identificabili come credibili sostenitori delle loro rivendicazioni. Quando si parla di crisi di rappresentanza del mondo del lavoro non si può non fare riferimento all'incapacità di rappresentare per molto tempo il lavoro e i lavoratori autonomi. Oggi è un dovere per le istituzioni del nostro Paese occuparsi di una categoria di lavoratori che ha bisogno di nuove norme di protezione e di tutela, oggi deboli o, per alcuni versi, assenti. assenti. L'Italia è tra i Paesi quello con il più alto numero di lavoratori autonomi: oltre il 26

alla nostra, ma ritengo che ciò sia la conseguenza della drammatica crisi economica in cui ancora versa quel Paese e della perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro subordinato negli ultimi anni. L'alto numero di lavoratori autonomi nel nostro Paese ci consente però di porre in premessa una domanda: si tratta sempre di lavoro naturalmente autonomo o spesso si tratta di forme di lavoro sostanzialmente subordinato ma mascherato da lavoro autonomo? Perché, se è vera la seconda ipotesi (e noi sappiamo che è vera), affrontando questo disegno di legge, dobbiamo capire come le nuove norme possano scoraggiare quelle forme distorsive del lavoro autonomo vero e proprio. Parti dell'opposizione ritengono che questo disegno di legge incoraggi il lavoro "mascherato". Io penso, invece, che le nuove norme limitino l'utilizzo di questi rapporti per finalità distorsive. Lo fa innanzitutto quando, all'articolo 3, si definiscono abusive e prive d'effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso. Uno degli aspetti più positivi del disegno di legge mi sembra quello di porsi l'obiettivo di costruire per i lavoratori autonomi finalmente un sistema di garanzie e tutele (un aggiornamento del nostro *welfare*) capace di dare risposte alle esigenze di questi lavoratori che oggi non sempre hanno. Lo fa all'articolo 6, quando delega il Governo ad approvare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con la finalità di abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione destinate innanzitutto «agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà». Lo fa, ad esempio, anche prevedendo che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Ancora, l'articolo 12, introduce una norma richiesta da tempo, in particolare delle lavoratrici autonome: si prevede che l'indennità di maternità spettante per i due mesi precedenti al parto e per i tre mesi successivi, venga riconosciuta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Importantissimo è poi, l'articolo 13: «La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno Io avrei preferito che la norma si fermasse a questo principio ma purtroppo - almeno a mio parere - continua ad affermare: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente». Sempre in tema di maternità mi sembra importante la disposizione che prevede la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma da parte dei familiari della stessa. È prevista, tra l'altro, la possibilità di copresenza della lavoratrice e del suo sostituto. formalizza in maniera molto chiara il fatto che la collaborazione si intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. un provvedimento importante e richiesto. Avviandomi alle conclusioni, il secondo argomento affrontato dal provvedimento oggi in discussione, quello inerente il lavoro agile, rappresenta una opportunità di migliorare la gestione del contratto di lavoro, non rappresentando una tipologia contrattuale a sé stante.

infatti che sia indispensabile raggiungere un accordo formale tra le parti, tra datore di lavoro e lavoratore. In particolare, con il lavoro agile si concretizza la possibilità di incrementare la produttività e di agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. è quindi un provvedimento importante, atteso da anni da un mondo che ha bisogno di maggiore attenzione. Noi oggi lo facciamo, dando a quel mondo l'attenzione

nella quale il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo, come quello di chiunque tragga dalla propria professione e dalla propria il necessario per il proprio sostentamento, ha alcune esigenze di sicurezza. Esigenze che, in questo caso, non possono essere soddisfatte all'interno del contratto di lavoro, ma possono e devono essere soddisfatte nell'ambito del rapporto previdenziale. Si riconosce che anche il lavoro autonomo, come quello di qualsiasi altro operatore nel tessuto produttivo, può soffrire di abusi di posizione dominante dominante a situazioni di dipendenza economica nei confronti del committente, da cui derivano distorsioni contrattuali che devono essere corrette.

È importante anche la seconda parte del disegno di legge, che intende promuovere l'area del lavoro subordinato che più si avvicina

al caso cioè in cui, nell'ambito della giornata, della settimana, o del mese di prestazione lavorativa, il datore di lavoro e il prestatore si accordano perché la prestazione stessa possa svolgersi

Tuttavia, a proposito di questa parte del disegno di legge, credo che in relazione ad alcuni aspetti del provvedimento

sul punto che non si preserva l'agilità se l'accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui. Va bene l'obbligo di stipulare l'accordo in forma scritta, ma se si impone che l'atto scritto definisca anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (articolo 16), piccole e medie ad avvalersi di un consulente. Noi vogliamo invece che il lavoro agile sia una forma di lavoro, un modo di essere del lavoro subordinato, direttamente direttamente e facilmente accessibile anche da parte della piccola e media impresa, senza necessità di una formulazione che implichi la consulenza e quindi un costo aggiuntivo. contare che il dover specificare le forme dell'esercizio del potere direttivo presenta il rischio di un aumento del contenzioso giudiziale.

al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori - sono dunque ben due i destinatari di questo adempimento con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo che nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile - che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo di lavoro consiste in un'attività svolta mediante *computer* collegato a distanza con l'organizzazione aziendale: dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria o dove si preferisce, è francamente non apprezzabile. Se così è, mi chiedo se non sia il caso di apportare al testo quell'emendamento che - vorrei ricordare - in Commissione

Esso prevede che questo obbligo si imponga là dove ci sia uno specifico rischio aggiuntivo; quindi non in qualsiasi caso, ma solo in quei casi in cui per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, sussista un rischio aggiuntivo Dobbiamo stare attenti, nel voltare pagina e nell'inaugurare questa che non credo sia un eccesso di enfasi definire "nuova era del nostro diritto del lavoro", a non cadere in un errore che ha caratterizzato il diritto del lavoro della vecchia stagione. vecchia stagione. Noi non perdiamo occasione per promettere agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili. Ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iperregolazione e dell'imposizione di adempimenti che non non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo. La comparazione, nel panorama internazionale, non offre alcun caso in cui questa forma nuova del lavoro del XXI secolo sia appesantita da un obbligo di duplice comunicazione scritta al lavoratore e al rappresentante sindacale di un documento su rischi che non siano rischi specifici, che devono essere come tali individuati e segnalati. Ecco, aspetto; siamo qui per discutere di questo disegno di legge e non credo che una piccola correzione possa compromettere l'*iter*, che spero rapido, di questo provvedimento, che è ora solo in prima lettura. comunque ottimo il lavoro che è stato fatto in Commissione, e non solo dalla maggioranza, perché abbiamo anche accolto importanti contributi della minoranza per il miglioramento del provvedimento. Chiedo che anche il Governo valuti questi aspetti, per evitare che il lavoro agile di domani sia un po' meno agile di quello che potrebbe essere. **Saluto l'onorevole Gerardo Amarilla De Nicola, presidente della Camera dei rappresentanti dell'Uruguay. La ringrazio, benvenuto al Senato della Repubblica italiana. Grazie Presidente, oggi il disegno di legge n. 2233 lavoro autonomo e lavoro agile; sinceramente leggendo "autonomo e agile" ho associato la cosa a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare del centro destra e del centro sinistra! Ritrova nella parola agile (cioè che si muove con elasticità e sveltezza), ciò che oggi meglio vi caratterizza!

mentre l'Inps lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro *Jobs Act* che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento di licenziamenti! Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le assunzioni a tempo indeterminato crollano le assunzioni come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti "per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo". I dati resi pubblici dall'Inps parlano chiaro: in due anni i licenziamenti sono passati da 35 a 46 mila, il 31 per cento in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale governo Renzi che, abolendo l'articolo 18, ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta.

L'insicurezza galoppa, e continua a crescere senza freni il ricorso ai voucher che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura; il loro *boom* conta un utilizzo rispetto all'anno scorso di un + 80 cento, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili. Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso... del -88 per cento!!!! Un successone!!!! II saldo sui contratti stabili dei primi otto mesi del 2016 è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale: da lì in poi in Europa ricominciano i numeri positivi, in Italia no. Insomma si stava meglio quando si stava peggio. Alla luce di questi dati non idilliaci per i cittadini permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando dì inventarsi attività in proprio e in autonomia, sempre più italiani cercano rifugio all'estero! Siamo sull'ordine dei 100.000 all'anno!

E oggi ci ritroviamo in questa Aula a discutere su un disegno di legge che è stato definito anche come il "*Jobs Act* del lavoro autonomo". Se le premesse sono quelle di cui sopra non c'è da stare allegri. Già il primo *Jobs Act* è stato una *débàcle*; con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere il Governo? Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse: il lavoro autonomo e il lavoro agile.

per onestà dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente. Questo lo diciamo perché quando c'è una cosa buona non ci tiriamo mai indietro. Anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele per il lavoratore. Il disegno di legge si pone poi l'obiettivo dì intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definita di lavoro agile o *smart working*; ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare il lavoratore. Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, che non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche a chi lavora in azienda, introducendo un'ulteriore flessibilità

Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo e ancora... il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, regolato,

qualche piccola concessione che troviamo in questo disegno di legge ma che non aiuterà il Paese a ripartire. Che dire! Chiuderei il mio intervento con una frase di un mio conterraneo il toscano Gino Bartali

Benvenute e benvenuti al Senato e in bocca al lupo per il vostro percorso di carriera.

delle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il cosiddetto lavoro agile, come previsto dal disegno di molto importante per il lavoro autonomo in quanto detta norme di protezione rilevanti per questo specifico settore, che spesso è stato dimenticato dal legislatore nazionale. Rappresenta, infatti, un atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale e ne valorizza il ruolo centrale nell'economia del nostro Paese. L'obiettivo principale è costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro, costituire un punto di riferimento di qualsiasi persona che voglia diventare un professionista investendo sulle proprie capacità e competenze. Detto questo, l'approvazione del provvedimento rappresenta un momento importante anche nel processo di ammodernamento dell'Italia, un processo promosso già dai precedenti Governi.

pari a quattro milioni di persone. Essi da tempo richiedevano una serie di interventi per essere maggiormente competitivi nel mercato europeo, a beneficio della concorrenza e della ripresa. tutti coloro non organizzati in ordini e collegi: se si considerano solo i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, si è registrata tra il 2009 e il 2013 una crescita pari al 19,1 Le nuove professioni registrano profondi cambiamenti e le nuove tendenze presenti nella società e in un mondo sempre in divenire. Oggi le imprese, per competere sul mercato globale, necessitano di servizi innovativi e ad alta specializzazione che vengono loro forniti dai nuovi professionisti in grado di trasformare i bisogni della società in virtù delle loro capacità e competenze. Su questo settore non siamo all'anno zero. È bene ricordare che il presente Governo è già intervenuto con il *jobs act* realizzando un'importante opera di pulizia delle finte partite IVA e false collaborazioni, ridefinendo dallo scorso 1° gennaio il perimetro della subordinazione, prevedendo la stabilizzazione dei rapporti autonomi fasulli e punendo con sanzioni economiche le violazioni. Ricordiamoci anche di questo. Fatto questo quadro in premessa, il provvedimento in esame rappresenta la seconda fase della riforma del lavoro e ha l'obiettivo di valorizzare l'autentico lavoro autonomo attraverso interventi normativi, innovativi e organici di riconoscere e utilizzare al meglio le energie positive di molti liberi professionisti in un quadro regolatorio omogeneo e coerente ai bisogni e alle aspettative di questi lavoratori.

una misura proposta del PD accolta in Commissione. Mi riferisco all'estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata e per entrambi i genitori il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino; all'esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e

la misura approvata, su cui avevo presentato una specifica proposta emendativa, che prevede per le lavoratrici e i lavoratori che devono sottoporsi a trattamenti oncologici e, dunque, sono inabili anche per un lungo periodo il riconoscimento della degenza ospedaliera, come per altre patologie gravi e invalidanti. Stiamo parlando, oltre che dei malati oncologici, anche di chi soffre di diabete, di sclerosi, di morbo di Parkinson, di insufficienze cardiache, respiratorie e renali, di Alzheimer, di fibrosi cistica e di altro ancora. È per questo, e per le altre misure, che ho detto che questa riforma del lavoro autonomo è importante. Essa estende una serie di diritti anche a chi prima non li aveva. Passo ora all'analisi del cosiddetto lavoro agile. Quello che viene chiamato anche *smart working* è un processo davvero di profondo cambiamento che riguarda l'organizzazione nel suo complesso, il modo di impostare il lavoro e di gestire anche le relazioni. Non è una forma di *welfare* aziendale e neppure un telelavoro che consente di far lavorare nelle mura domestiche una volta alla settimana. È una nuova filosofia aziendale, che restituisce flessibilità e autonomia alle persone nelle proprie scelte lavorative. Per comprendere l'attenzione verso questo nuovo modello, che è già praticato da molte multinazionali e da diverse aziende di grande importanza ed entità, occorre considerare alcuni punti critici del sistema di organizzazione del lavoro italiano. Abbiamo un *gap* di produttività - ci rivelano - inferiore rispetto alla media media europea, un *engagement* di lavoratori, rispetto alle loro attività, limitato. Secondo una rivelazione recentissima, in Italia le persone motivate rispetto al proprio lavoro sono solo il 59 per cento, al di sotto di altri Paesi, bisogna pensare anche di rimotivare i lavoratori. Non poche persone - abbiamo scoperto - preferiscono lavorare per obiettivi, per fasi, per cicli, ed essere valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri quali l'ora di lavoro, la presenza fisica nei locali aziendali, lo spazio. La mobilità e il cambiamento di occupazione sono più visti non in negativo, ma anzi come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

e si mantiene alto il tasso di abbandono dopo la maternità: il 22 per cento delle madri lascia il lavoro entro il compimento del secondo anno del primo figlio. Quindi, ripensare il modello di lavoro che segua le logiche dello *smart working* ha aspetti positivi e incoraggia il lavoratore a essere motivato. Può, poi, influire su chi si muove, sull'inquinamento, motivo per cui molte amministrazioni pubbliche locali hanno avviato iniziative di sensibilizzazione verso aziende e organizzazioni territoriali.

percorrono tanti chilometri in media durante la giornata, con 33 giornate lavorative annue. Consentendo loro di lavorare da casa o in ufficio, ma fuori dagli orari di punta, si risparmierebbero giornate lavorative perse nel traffico; si avrebbe meno stress e un aumento di produttività lavorativa. Quindi, anche Quindi, anche in questo caso direi che è ora di cambiare. *Smart working* significa ridefinire il lavoro in maniera più efficiente e agile, ridando alle persone la facoltà di decidere dove e quando lavorare, ovviamente in cambio di migliori risultati per l'organizzazione, le persone e la collettività.

non può utilizzare normalmente i mezzi pubblici o privati. Per tali soggetti diventa prioritario poter accedere a formule e modalità organizzative del lavoro che consentano la più ampia libertà Una cornice normativa sarà certamente di grande aiuto se accompagnata da idonei incentivi (ricordo il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) e da una contrattazione collettiva di sostegno. Per questi motivi, ritengo che il provvedimento in esame debba essere assolutamente

certo il pregio di introdurre significative misure a favore di categorie particolarmente esposte, a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale. di una misura che guarda anche - io spero soprattutto - alle giovani generazioni, a coloro che sono impiegati nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione: tutte categorie che provano ad affacciarsi al mondo del lavoro con una voglia di fare e, per questo, non possono essere mortificate, come spesso succede. Il grave problema del recupero crediti soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, l'assenza di tutele in caso di malattia o maternità, la difficoltà di accesso al credito,

Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore che è vasto e particolarmente eterogeneo e articolato. Tuttavia, esso ci convince anche nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l'obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all'efficienza e ai risultati. di un importante passo in avanti anche per alcune professioni che necessitano non della presenza fisica, ma di uno spazio virtuale in costante connessione, dove chi lavora

Il primo ordine del giorno è volto a impegnare il Governo ad approfondire la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale, ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). A nostro avviso, anche al fine di avere un quadro molto più chiaro delle situazioni contributive dei vari soggetti, è necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata. Il secondo intervento, in virtù di quanto introdotto con l'articolo 16 di questo provvedimento, riguarda la necessità di dare un'interpretazione autentica delle norme relative alle indennità per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito. Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova. ringrazio la Commissione e ringrazio che questo provvedimento sia stato calendarizzato in Aula e spero che

*(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. È nelle premesse del provvedimento come negli ultimi due decenni il sistema produttivo italiano sia stato caratterizzato da profonde trasformazioni. La composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, vedendo crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma non solo autonoma ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto "atipiche". Allo stesso tempo, i dati ISTAT mostrano come, in questi anni, le stesse forme di lavoro autonomo o soggette a contrattualizzazione "atipica" hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire un corpo sociale a sé, che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Anche sotto il profilo della precarietà, i lavoratori autonomi e "atipici" hanno mostrato una condizione di ulteriore instabilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione in sé quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele. Questo disegno di legge interviene, quindi, per restituire ai lavoratori autonomi una rete di tutele e diritti che mancava, un passo che era atteso e necessario e va riconosciuto l'impegno del Governo e del Parlamento, e quindi del nostro Senato, nel portare avanti questo provvedimento. Abbiamo svolto molto lavoro in Commissione, con audizioni e confronti. Le misure sono state anticipate dagli altri interventi e dal relatore. Oggi utilizzerò il tempo che mi è concesso per riprendere due argomenti che, nell'ambito del tema lavoro autonomo e atipico dovranno essere quanto prima affrontati proprio per rafforzare il provvedimento che oggi discutiamo. La nostra Costituzione, all'articolo 36, stabilisce che: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», sottolineando l'importanza fondamentale del lavoro, come chiave della crescita sociale ed economica del nostro Paese. Il lavoro duro delle precedenti generazioni ha permesso al Paese di rialzarsi e crescere nell'immediato dopoguerra fino a essere tra le prime economie mondiali. Ma tale impegno sarebbe stato vano se non fosse stato accompagnato dalle garanzie sociali, acquisite nel tempo, che hanno permesso - ad esempio - di acquistare le case di famiglia e di maturare quelle pensioni che oggi sostengono moltissimi giovani, figli e nipoti, costretti a barcamenarsi con lavori precari, spesso mascherati da lavoro autonomo ma subordinati di fatto, genericamente sottopagati, almeno fino all'approvazione di questo disegno di legge, e privi delle tutele e dei diritti che, a fatica, negli anni erano stati conquistati e della dignità che ogni lavoro onesto dovrebbe dovrebbe suscitare in chi lo svolge. Ricordo - ad esempio - l'esperienza e la protesta dei fattorini di Foodora a Torino. Negli ultimi anni è cresciuto in modo pericolosamente esponenziale il numero dei lavoratori che sfuggono alle maglie della contrattazione collettiva e hanno redditi al di sotto della soglia di povertà. La povertà è, di fatto, aumentata in senso assoluto. Sarebbe quindi necessario mettere in campo una misura - penso all'equo compenso o al salario minimo orario per tutte quelle categorie di lavoratori per le quali sia assente un contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo scopo è garantire un livello di reddito per i lavoratori, utile a garantire per gli stessi un tenore di vita dignitosa, mantenendo, nella loro partecipazione al lavoro, una concorrenza leale tra loro e i datori di lavoro per evitare il cosiddetto *dumping sociale*. E ciò è necessario proprio al fine di promuovere la coesione sociale e favorire la redistribuzione del reddito.

L'esistenza di una misura a garanzia del compenso avrà un effetto positivo a lungo termine sul livello di occupazione, incoraggiando i lavoratori a investire nel proprio posto di lavoro, le aziende a promuovere formazione continua e guadagni di produttività, e lo Stato a formare i suoi cittadini. Le misure contro la precarietà e la disoccupazione sulle quali siamo impegnati hanno bisogno di completarsi con la realizzazione di un efficace e sistemico programma di "orientamento al lavoro". Il mondo delle professioni - i cui rappresentanti abbiamo avuto modo di audire - è vario e ricco di esperienze e professionalità e anche di opportunità. mettere a disposizione degli studenti che stanno completando i loro cicli di studio e dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, oltre che la corretta formazione, una corretta e completa informazione sui percorsi professionali disponibili sul proprio territorio, offrendo a ognuno la possibilità di valutare non solo i percorsi più vicini alle proprie inclinazioni, ma anche quelli reciprocamente più utili e soddisfacenti, e non solo per il lavoratore, ma anche nell'interesse economico e sociale del Paese, tenendo conto dei processi di evoluzione del mercato del lavoro stesso. stesso. Molte offerte professionali, infatti, restano inevase e di fatto sconosciute, mentre per altre professioni più convenzionali le richieste superano di gran lunga la loro naturale offerta generata dal mercato. I professionisti in eccesso in un determinato settore si trovano, dunque, a dover accettare lavori inferiori o eccessivamente distanti alla loro formazione e aspettativa, incrementando, quindi, oltre alla precarietà, frustrazione e disaffezione sociale. Si parla molto di "buone pratiche": in questo settore un esempio eccellente da seguire ce lo offre la Germania, il cui programma di orientamento al lavoro va incontro a studenti e famiglie, prevedendo, fra le numerose misure, degli incontri annuali obbligatori con le classi in "uscita" di ogni istituto e offre loro un contatto costante con i consulenti. in esame si compie un primo passo, con la previsione dello sportello per le professioni, all'interno dei centri per l'impiego. Infatti, una delle misure più strategiche sul lungo periodo del *jobs act* è l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro cui statuto richiama proprio la dignità costituzionale che è propria dell'Agenzia, in quanto specificatamente volta a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all'ANPAL la responsabilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È su questo punto, dunque, che Presidente, la discussione di oggi ha come oggetto una questione delicata, urgente e prioritaria, che ci impone un'analisi oculata dei provvedimenti che ci giungono dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato e ci obbliga ad accantonare le diatribe e lo scontro politico. Noi, come opposizione, siamo pronti a farlo. Mi auguro che la maggioranza sia altrettanto pronta e disponibile ad abbandonare quell'atteggiamento che, in molte occasioni, ha permesso non un confronto, un dialogo, ma solo imposizioni a colpi di voti di fiducia. L'impianto generale di entrambi i disegni di legge rappresenta un tentativo, naturalmente correggibile in alcuni aspetti, di porre fine alle disparità nel mercato del lavoro, cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA e dei liberi professionisti. Sappiamo che il mondo del lavoro e l'approccio verso il mercato del lavoro sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di venti o di dieci anni fa e le leggi devono adattarsi. La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostra l'aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti diritti e garanzie. Cari colleghi, il lavoratore è forte quando è forte il mercato. E uno degli aspetti interessanti di questo disegno di legge è forse quello della creazione di uno sportello di intermediazione che raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornirà le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno richiesta. Occorre, però, porre in essere tutte quelle sinergie operative per far sì che il meccanismo delle funzioni non si traduca nell'ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze di quanti si affacciano al mondo del lavoro. Su questo, come in molti altri aspetti, abbiamo visto con favore, nel corso della discussione in Commissione lavoro, accolti alcuni nostri emendamenti. Altri sono stati poi recepiti dal relatore, che li ha evidentemente considerati un apporto positivo al testo in esame. Parlo - ad esempio - del richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, esperibile anche attraverso gli organismi abilitati o, ancora, di ampliare il perimetro dello sportello prima citato, anche agli organismi autorizzati all'intermediazione. In quest'ultimo caso però non si è ritenuto - o forse non si è voluto - accogliere un nostro emendamento che integrava la norma con una precisa tipologia di enti che già svolgono questa funzione. Mi riferisco ai patronati che, per la loro provata esperienza nel campo previdenziale e lavorativo, la loro presenza capillare in tutto il territorio nazionale, la professionalità e la qualificazione del loro personale possono espletare tutte le procedure indicate nella norma. Occorre infine sottolineare che i centri per l'impiego sono oggi sottodimensionati e in enorme difficoltà nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni. L'estensione della norma agli istituti di patronato rientrerebbe nelle "attività diverse" riconosciute dal Ministero del lavoro e avrebbe l'effetto di migliorare il servizio offerto ai cittadini. Ma sappiamo che il Governo - salvo repentini ripensamenti, in questo periodo molto frequenti motivati da necessità referendarie - da tempo ha deciso di eliminare dal suo vocabolario la parola concertazione e con essa tutto quanto a essa riferibile, dunque anche i patronati che in molti casi, ma non per tutti, sono emanazione diretta delle organizzazioni sindacali. Dovremmo, altresì, riflettere sulle tutele relative al rapporto con il committente. Le clausole inserite mirano a salvaguardare il lavoratore autonomo da clausole e condotte abusive da parte del committente. Verranno considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o di recedere senza congruo preavviso, o saranno considerate abusive quelle clausole mediante le quali le parti concorderanno i termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su quest'ultimo punto è doveroso precisare che dovremmo estendere l'applicazione di questa clausola anche alle pubbliche amministrazioni che, nonostante il limite di trenta giorni, spesso si contraddistinguono per tempi di pagamento estremamente proprio "suicidio economico" sia del libero professionista sia delle piccole e medie imprese. Se lo Stato impone che le regole vengano rispettate nell'interesse e tutela dei lavoratori, dovrebbe essere il primo a rispettarle. Tornando alle clausole e condotte abusive, riteniamo alquanto rischioso affidare agli accordi tra azienda e lavoratore l'individuazione delle condotte che danno luogo a sanzioni rinviando ai contratti collettivi, e a tal proposito abbiamo presentato apposito emendamento. Un altro aspetto che ci preoccupa è quello contenuto all'articolo 5 della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche. Ebbene, la norma nel complesso parla di "atti pubblici" al comma 1, che sono quelli posti in essere secondo il dispositivo dell'articolo 2699 del codice civile, e di atti delle pubbliche amministrazioni alla lettera del criterio di delega, che ovviamente riguarda ogni atto da svolto dalle pubbliche amministrazioni. Andrebbe quindi meglio chiarito il perimetro della norma, anche legando la rimessione di tali atti sulla base di criteri non solo di terzietà, ma anche di competenza professionale specifica. In tal senso il nostro Gruppo ha presentato degli emendamenti. In ogni caso, riteniamo che l'impianto generale dei due disegni di legge in discussione sia positivo, salvo per il fatto che - come è ormai prassi consolidata di questo Governo - si ricorre alla solita previsione di norme di delega - ve ne sono ben tre differenti - un modo discutibile per rinviare la soluzione del problema all'emanazione di futuri decreti legislativi che - come tutti sanno - prevedono solo un parere, non vincolante, da parte del Parlamento. Rimane però un provvedimento che potrebbe snaturare la vera natura delle partite IVA. È giusto prevedere garanzie e diritti ai lavoratori autonomi, ma occorre fare attenzione a non imbrigliare il lavoro autonomo nelle regole del lavoro dipendente.

del Partito Democratico e mi rendo conto che la realtà è un po' diversa. Provo a riassumere: poiché il lavoro autonomo è stato snaturato, poiché la difficoltà del momento ha fatto sì che tante imprese

per minore assenteismo. Non esiste l'assenteismo nel lavoro autonomo, perché assenteismo vuol dire non lavorare, il che vuol dire non mangiare. Sarebbe un settore da mettere sotto il riflettore e assumere come modello emblematico per tutto il resto.

A noi è piaciuto perfino l'inserimento della norma anti-furbaggine: non ti do denaro perché mi racconti che hai perso mercato, perché è

che gli autonomi, volenti o nolenti, abbiano un socio (in questo caso lo Stato italiano) che li spreme per quasi due terzi (e a volte anche di più) del reddito che riescono a produrre. Vorrei parlare ancora di chi vuole intraprendere lavori autonomi.

possiamo spendere deriva proprio da questi lavoratori. Auspico inoltre che non si senta più dire in quest'Aula che il settore va aiutato perché tanti dipendenti camuffati devono diventare degli autonomi: o aiutiamo i lavoratori autonomi o continuiamo a fare altre cose.

Signor Presidente, colleghi, vi sottopongo un ennesimo caso di incoerenza politica tra quello che si dichiara e quello che poi si compie.

È stranamente fermo, perché da più di un anno tutta la politica dice di essere d'accordo su questo provvedimento, che è positivo e va portato al più presto a buon fine.

troppi poteri e troppo spesso li utilizza male. Nonostante la politica da un anno dica che è importante dotarsi di una norma più trasparente ed efficace, la discussione, da marzo ad oggi, non si è mossa di un passo. E questa, cari colleghi, è l'ennesima dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, che non è la Costituzione che rallenta il processo normativo, ma è la volontà della maggioranza. Mi rivolgo agli italiani che ci guardano in televisione: è la maggioranza che decide la calendarizzazione nei lavori di Commissione e in Aula. Queste sono le regole ed è giusto rispettarle, ma è la maggioranza che si assume la responsabilità di che cosa viene portato in discussione e che cosa non viene portato in discussione. Questo è un provvedimento che tutti da un anno dicono di voler portare a termine; allora portiamolo a termine. Quindi il mio appello non è alla Costituzione, che va benissimo così, è a posto così; il mio appello è alla maggioranza: agite coerentemente con le vostre dichiarazioni. Signor Presidente, colleghi, la problematica che come Italia dei Valori vogliamo porre all'attenzione si incentra sulla legittimità di una serie di contratti stipulati dalla società Poste italiane, nella persona della dottoressa Barbara Poggiali, con soggetti esterni rispetto alle risorse presenti in azienda per l'espletamento di attività che potevano e dovevano essere svolte da personale dipendente dell'azienda stessa. In altri termini, ci si chiede come si possa rendere un'attività ordinaria, nel senso di rientrare nelle competenze del personale dirigenziale e manageriale già presente nella società Poste italiane, in attività straordinaria. Vi spiego meglio. La dottoressa Barbara Poggiali attualmente, con decorrenza immediata dal 30 settembre 2014, ricopre la funzione di direttore *marketing* strategico della società Poste italiane. Dai documenti contabili aziendali sembrerebbe emergere come dall'annualità 2014, precisamente dal mese di dicembre, le spese effettuate al fine di usufruire della consulenza della società The

i prezzi netti di acquisto per progetti o consulenza o supporti operativi - successivamente al mese di settembre 2014, sembrerebbero arrivare sino ad oltre un milione di euro per singolo progetto. Nella sostanza, si giunge nell'arco di quasi un biennio (dicembre 2014-settembre 2016) allo stanziamento di oltre 12 milioni di euro. Ne emerge un frazionamento di incarichi (circa 12 nel 2015), verso la medesima società di consulenza, i quali restano, a buon bisogno, contenuti al di sotto di un milione di euro e, pertanto, con frazionamento di spesa ed in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia di gara per l'affidamento di servizi e con divieto, dunque, di procedere ad affidamento diretto. Ed ancora, ne emerge l'assenza di qualsiasi indicazione circa la necessità di specifiche competenze professionali e comunque di una verifica sulla presenza di figure professionali interne e in servizio idonee allo svolgimento degli incarichi esternalizzati. Occorrerebbe accertare la carenza nella società Poste italiane (nel settore *marketing* strategico), sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, delle competenze professionali idonee a svolgere i servizi conferiti di volta in volta alla Boston consulting group. Le società partecipate da pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di conferire incarichi professionali nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come si impongono esigenze di contenimento della spesa pubblica e la garanzia della trasparenza e della meritocrazia nell'affidamento di incarichi professionali. Occorre infatti evitare che incarichi dalla durata pluriennale, aventi ad oggetto prestazioni di tipo non specialistico, nascondano fini clientelari, unitamente all'intento di assicurare la massima pubblicità per consentire il controllo popolare sull'utilizzo del pubblico denaro. Poiché il tempo a mia disposizione

Frequenti negli ultimi mesi, infatti, erano state le notizie apparse sulla stampa in merito all'insistenza, in queste zone, di fenomeni di sfruttamento di lavoratori agricoli indiani della cosiddetta comunità sikh.

Nel corso dell'ispezione è emerso un quadro grave circa le condizioni di lavoro di oltre cento braccianti di nazionalità indiana, caratterizzato dall'omissione di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dall'audizione di alcuni lavoratori è risultato che questi venivano costretti spesso a lavorare undici-dodici ore al giorno, per una paga di circa 3 euro l'ora, e sottoposti a vessazioni e mortificazioni, in un clima di paura, divenendo finanche oggetto di intermediazione illecita da parte di caporali. A seguito di tale ispezione, la procura della Repubblica di Latina ha proceduto per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e, in data lunedì 24 ottobre scorso, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cittadino indiano accusato di aver effettuato caporalato ai danni dei propri connazionali. Si tratta di un importante sviluppo processuale, che conferma l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, grazie al prezioso impegno - me lo faccia dire, signor Presidente - dei componenti della stessa, dei dirigenti e dei funzionari, della segreteria, dei carabinieri e dei consulenti

con attenzione alla tutela delle vittime, è possibile accertare i fatti di caporalato e contrastare efficacemente la piaga dello sfruttamento del lavoro. Ora si deve vigilare sull'applicazione della nuova legge, che ha riformato il reato estendendo l'incriminazione per intermediazione di manodopera

prendono sempre più il sopravvento e cercano di imporsi anche nei confronti delle istituzioni. Nel caso specifico questa mattina, davanti al comune di Tradate, è stata inscenata l'ennesima manifestazione da parte di un nutrito gruppo di richiedenti asilo presenti presso la la stessa cittadina, con l'obiettivo di ottenere il rilascio della carta d'identità. Ho avuto modo di approfondire in giornata con il prefetto le circostanze che hanno portato costoro ad avere questa pretesa ed è emerso uno scenario molto preciso. Una buona parte dei richiedenti, nel caso specifico, ha avuto già un diniego del riconoscimento dello *status* di profugo. Ciò determina chiaramente l'avvio di un percorso ulteriormente grave. Infatti, la richiesta del riconoscimento della residenza e, nel caso specifico, l'ottenimento della carta d'identità, pur in presenza di un diniego cui è stato opposto ricorso presso il tribunale, significa che costoro hanno colto una debolezza da parte del sistema italiano. Signor Presidente, non voglio sottolineare cosa significa avere in circolazione migliaia o decine di migliaia di carte di identità, in mano a gente che oggettivamente non ha alcun diritto di essere presente come profugo o che sia riconosciuta come avente diritto alla protezione sussidiaria sul nostro territorio nazionale. Il prefetto assicura che, nel momento in cui costoro dovessero avere in mano un foglio di espulsione, i documenti verrebbero ritirati. Sfido chiunque a immaginare come possano essere ritirate queste carte d'identità una volta rilasciate. Invece, se questa circostanza non verrà fermata, avremo in circolazione sul territorio nazionale - e voglio sperare non oltre - carte di identità legalmente rilasciate dai nostri uffici di stato civile; con quale uso e con quali rischi? Questo è un vero e serio problema che pongo. Credo che il legislatore (in questo caso, il Governo) debba prendere in seria considerazione questo fatto.

Grazie